per noi dell'Italia dei Valori questo decreto milleproroghe oggi in discussione in Aula ha almeno tre evidenti e dannose anomalie. La prima è che oggi se ne parla come se si trattasse di uno dei vari adempimenti che l'esame del bilancio dello Stato sottopone annualmente al Parlamento, in realtà questo strumento speciale, che fu inaugurato nel 2005 dall'allora Governo Berlusconi per far fronte entro la fine dell'anno alle questioni più urgenti, fatto trasformato in una procedura che, sia per i contenuti proposti, o meglio, imposti da questo Governo, sia per la ipertrofia abnorme di proposte emendative da parte di questa maggioranza (che nulla hanno a che vedere con il carattere dell'urgenza o della proroga e che avrebbero meritato tutt'altro approfondimento, e lo vedremo

necessarie di politica economica per il nostro Paese. La seconda anomalia è che anche questa volta il Governo non ha rinunciato ai suoi soliti proclami propagandistici nel titolare l'ultima parte del decreto «proroga di interventi di sostegno alle imprese e alle famiglie». Non c'è bisogno di scomodare le grandi categorie del pensiero economico per capire che non c'è niente di tutto ciò. Una prima smentita viene dalle modalità di copertura finanziaria individuate; ne cito solo alcune, due del Governo e una della maggioranza. In termini di saldo netto da finanziare, è prevista una copertura in questo decreto per 93 milioni mediante l'utilizzo di una quota delle risorse iscritte presso la contabilità speciale relativa a rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta: per capirci, sono proprio i crediti che vanno alle imprese. Il Governo aveva già modificato la norma con un tetto di spesa tipo *click day*: chi arriva per primo prende tutto, e i primi sono arrivati entro 60 secondi. Nella finanziaria 2011 il Governo poi intervenuto con il solito tappabuchi, con crediti di imposta per un totale soltanto di 100 milioni finalizzati ad attività di ricerca e sviluppo affidate dalle imprese ad università o enti pubblici; con decreti ministeriali si doveva poi decidere quando, quanto e a chi attribuire queste risorse. non contenti di tutto questo, alle imprese fate slittare di un anno anche il diritto al rimborso maturato: questo è il sostegno che viene dato alle imprese. Non va meglio per il sostegno al reddito delle famiglie. Le tre misure più significative in materia di lavoro - la prima per il lavoro occasionale di tipo accessorio; la seconda con la proroga dell'intervento di equiparazione dei lavoratori qualificati sospesi e degli apprendisti ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali; la terza con la possibilità di adeguare le norme che disciplinano i fondi di solidarietà dei settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni - non presentano oneri aggiuntivi: neppure un euro in più. Non ne derivano ossia maggiori oneri, in quanto trovano applicazione nei limiti di risorse già previste per il 2011 a legislazione vigente. Peccato che in Italia uno degli ultimi monitoraggi del Ministero del lavoro stimi che gli ammortizzatori sociali non coprono più del 30 per cento dei disoccupati, con sussidi di varia natura; e gli altri? Si devono arrangiare da soli. Il terzo esempio. Mentre l'Unione europea ha già aperto un *dossier* con il rischio di infrazione per la proroga, contenuta nell'ultima finanziaria, del pagamento delle multe per le quote latte; mentre il commissario straordinario per le quote latte parla di un totale di 280 milioni che lo Stato deve recuperare; mentre il ministro Galan, di questo Governo, si appella al rispetto della legalità e dell'etica e tutte le associazioni - Coldiretti, CIA, Confagricoltura - gridano allo scandalo perché questa vicenda ci è già costata 1,7 miliardi di euro pagati dai contribuenti italiani, la maggioranza impegna, con un emendamento approvato, 30 milioni che vanno a copertura dell'ulteriore proroga delle multe per lo sforamento delle quote latte. E questi milioni da dove vengono? Vengono di fatto prelevati dai fondi per le politiche sociali, il diritto allo studio, la famiglia. E allora non dobbiamo meravigliarci se pensiamo alle risorse destinate a copertura del 5 per mille. Apparentemente - dico apparentemente - il milleproroghe reintegra la somma a 400 milioni. Ma l'onere aggiuntivo sul bilancio pubblico è di soli 200 milioni, e una quota pari a 100 milioni è destinata a interventi per la sclerosi laterale amiotrofica, anche se la legge di stabilità aveva già destinato 100 milioni a interventi per la SLA a titolo di fondo per i non autosufficienti. Così, con soli 100 milioni di euro, si potrà dire di non avere cancellato il Fondo per le non autosufficienze e di aver reintegrato il cinque per mille, anche se il primo di fatto è stato ridotto di 300 milioni ed il cinque per mille di fatto è stato tagliato di 100 milioni. Questo è un bell'esempio di finanza creativa. La terza anomalia che riscontriamo in questo decreto è che il sistema delle proroghe ad oltranza danneggia - e lo si è visto in più occasioni - qualsiasi possibilità di programmazione e serve a mascherare l'incapacità di questo Governo, che non è in grado di concepire riforme organiche, a lungo termine. signor rappresentante del Governo, è la proroga dell'articolo 6-*sexies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e la riprogrammazione unitaria delle risorse del quadro strategico nazionale, ossia delle modalità di impiego dei finanziamenti destinati originariamente a progetti cofinanziati dal bilancio comunitario. La relazione tecnica ci spiega perché. La proroga è volta a delineare un percorso celere e di maggiore certezza ai fini dell'attuazione del tanto annunciato, famigerato, Piano nazionale per il Sud. A distanza di quasi tre anni manca ancora un serio lavoro, di ricognizione prima e di elaborazione poi, delle risorse da destinare ad un progetto compiuto di sviluppo per il Paese e per il Mezzogiorno. Altro che piano per il Sud, altro che scossa all'economia! Ci troviamo di fronte, ancora una volta, al solito diversivo per distrarre l'attenzione dalle vicende giudiziarie e, diciamo anche, sentimentali del Capo del Governo. Per non parlare poi della programmazione sulla sanità. Con la proroga degli accreditamenti provvisori alle strutture private, con la possibilità di utilizzare le risorse *ex* articolo 20 per l'edilizia sanitaria non per una nuova programmazione ma per interventi già effettuati, e con l'ulteriore proroga del passaggio a regime ordinario dell'attività libero-professionale dei medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, già previsto nel 2007, di fatto avete smantellato una seria riprogrammazione sanitaria. Per non parlare di altre iniziative riformatrici ferme al palo ed ulteriormente prorogate per un'assenza totale di dialogo e di cooperazione interistituzionale tra Stato e Regioni.

milleproroghe. Tralasciamo per amor di Patria quelli rivolti ad alcune categorie di privilegiati, come la riduzione dell'anzianità di servizio per l'accesso alla qualifica dirigenziale a prefetto o l'allocazione di nuovo personale ai quattro dipartimenti dell'Amministrazione finanziaria, in un Paese come il nostro che ha chiesto al pubblico impiego il sacrificio del blocco del *turn over*, del blocco delle retribuzioni e degli scatti di anzianità. Mettiamo da parte il diverso metro di giudizio per la valutazione delle proroghe delle graduatorie concorsuali, per cui ad alcune si concede una protezione addirittura territoriale e ad altre, come quella dei vigili discontinui, neppure lo slittamento di un anno a costo zero per portare avanti quel percorso di stabilizzazione avviato con la finanziaria 2007 che poi è stato traumaticamente interrotto. Mettiamo da parte anche i criteri con cui vengono elargiti i contributi in questo decreto milleproroghe, come i 2 milioni di euro per il festival Verdi sopprimendo l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni, senza sapere che non è di poco conto che questo ufficio (l'UNAR), nato per volontà dell'Unione europea, insediato in tutti i Paesi europei e sostenuto da risorse comunitarie, avviato nel solo anno 2010 nei confronti di enti pubblici ben 790 segnalazioni di discriminazione, quasi tutte accolte dai tribunali; o il contributo di 200.000 euro per l'Associazione alleanze degli ospedali italiani nel mondo con fondi prelevati dalle risorse per la ricerca e l'assistenza ai malati oncologici (associazione certamente di pregio, come tante altre, anche se

per le emittenti radiotelevisive di alcune Regioni autonome. Noi, signor rappresentante del Governo, vogliamo richiamare la vostra attenzione su due aspetti trattati in questo decreto. Il primo è l'emergenza "fai da te", detta anche federalismo delle tasse: la logica federalista, cioè, nel nostro Paese vale anche in caso di disgrazia. Le Regioni colpite da una catastrofe, se non riescono a coprire le spese della ricostruzione, dovranno aumentare i tributi, le addizionali regionali, l'imposta regionale sulla benzina, e se le tasse non basteranno e si richiederà l'intervento del Fondo nazionale per la protezione civile, anche in questo caso il Fondo è da integrare con l'aumento delle aliquote sulla benzina. È questo un ulteriore passo indietro rispetto alle modalità con cui è stato trattato l'Abruzzo, per il quale si prevede sì una sospensione dei tributi per nove mesi, ma senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, come a dire che entro l'anno, se non interverranno altre proroghe caritatevoli o misericordiose, si dovrà pagare il pregresso e il nuovo. Il secondo aspetto, signor rappresentante del Governo, a sottolineare il disimpegno di questo Esecutivo in un settore così importante e delicato come quello dei servizi sociali, è l'intervento sulla povertà. Con questo decreto creiamo quasi una povertà di serie A e una di serie B, una povertà di città ed una di periferia. In questi ultimi due anni, i servizi sociali sono stati pesantemente tagliati da questo Governo, creando un panorama desolante, con il Fondo nazionale per le politiche sociali ridotto di un terzo, il Fondo per le politiche della famiglia ridotto a 51 milioni e il Fondo per la non autosufficienza quasi del tutto azzerato. Ebbene, il Ministro dell'economia nell'altro ramo del Parlamento ha stimato che il programma per la carta acquisti, la famosa, famigerata *social card*, tanto propagandata come risolutrice di molti problemi,

degli enti caritatevoli che operano nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. E le Regioni che non hanno Comuni con questo numero di abitanti? Continueranno ad avere quello che hanno avuto sinora, cioè poco o nulla. nulla. Queste, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, sono soltanto alcune considerazioni, di forte criticità

l'unica proroga che veramente pesa in questo decreto è quella delle difficoltà e dei problemi che gli italiani continuano ad avere e che non sono stati assolutamente affrontati o che non si è tentato di affrontare. Quindi, riteniamo che, se il Governo non ha avuto l'interesse o la capacità di affrontare questi problemi, almeno debba avere il coraggio

Presidente, signor Sottosegretario, colleghi relatori,

questo mosaico impazzito che è diventato il milleproroghe. Altri colleghi hanno detto assai bene cosa, nel corso del tempo, è successo a quello che si chiamò milleproroghe in altre stagioni. un testo, ma anche un ipertesto, un sottotesto, con metatesto, un'iperbole, una sineddoche, un ossimoro, un insieme di aporie; è un po' un dramma e un po' un melodramma. Vorrei che si scorresse di più l'articolato affinché non sfuggisse qua e là, nel *latinorum* dei tanti commi, quello che è accaduto alla cultura italiana. Quest'ultima è ridotta ad una mancia di 15 milioni di euro; ne occorrevano dieci volte di più per sanare un po' la situazione del cinema, della musica, del teatro, della danza e così via.

come al solito, del leone anche su quella strana vicenda del fondo del ministro Romani per la banda larga (come le "vacche di Mussolini"); sono due anni che girano quei milioni di euro e ora cadono forse su una banda larga

Vorrei dedicare la parte conclusiva del mio intervento, a proposito di editoria, ad un vero e proprio fatto inquietante del testo.

motivo: scadeva il 31 dicembre 2010 uno degli ultimi punti della normativa *antitrust* italiana (come sapete assai labile, certo non rigorista né rigorosa; non è un Paese calvinista); scadeva uno di quei pochi paletti *antitrust*, cioè il divieto, per chi ha più di una rete televisiva generalista terrestre, di acquisire giornali quotidiani. È accaduto che un nostro emendamento, ovviamente respinto, poneva l'ovvietà, ossia che quel termine scorresse ancora per qualche anno, diciamo almeno fino a compimento della famosa rivoluzione digitale. Avevamo stabilito il 2016, ma si poteva immaginare anche un anticipo, per dare una qualche cognizione di causa alla normativa così tribolata - usiamo un eufemismo - in questo sistema. Invece, in un decreto milleproroghe (vorrei che voi udiste bene: milleproroghe, cioè proroghe appunto dovevano essere) c'è un vero colpo di mano normativo e ordinamentale (come dicono i giuristi). Con questo testo cosa succede? Accade che il divieto (si fa per dire; le norme *antitrust* sono molto aggirate - come sappiamo - in Italia) non riguarda più seccamente, come era, chi ha più di una rete televisiva terrestre, ma improvvisamente chi ha più dell'8 per cento di quella strana

un gruppo che dà qualche fastidio al "partito azienda" che ha molti legami - com'è noto - con la Presidenza del Consiglio, cioè il gruppo Sky, che è oltre l'8 per cento. Pertanto Sky non può entrare in un gruppo editoriale. Non ho simpatie per nessuno; facendo questa attività, bisogna essere laicamente distanti.

mediatico-politica italiana e quindi guai se mette il naso nella stampa quotidiana. Naturalmente i dati che oggi emergono da numerosi organi di stampa su ciò che avviene nella compagine societaria del quotidiano fa pensare che quel limite dell'8 per cento sul SIC, essendo così labile, non impedirebbe da sé un eventuale interesse di Fininvest-Mediaset per l'entrata in questa compagine turbolenta del quotidiano «Il Corriere della Sera»: una vecchia ambizione del

Per chi è credente in quest'Aula, non creda con questo di non andare all'inferno: il peccato resta mortale e questo non vi salva.

Spiace però notare che alcuni colleghi abbiano sottolineato negativamente l'approvazione di molti emendamenti in Commissione: qualcuno ha parlato addirittura di stravolgimento. se dei circa 1.500 emendamenti presentati ne fossero stati approvati solo cinque o dieci, non si sarebbe potuto neanche immaginare di parlare di stravolgimento del testo; ma questo avrebbe significato non tenere conto delle proposte di tanti colleghi senatori. Credo che possiamo essere contenti di aver fatto delle modifiche anche importanti; anche importanti; naturalmente non tutte piaceranno a tutti, questo è nei meccanismi parlamentari, ma credo che sia stato un fatto positivo aver potuto considerare con attenzione tutte le tutte le questioni sollevate, dando ad alcune risposte soddisfacenti, ad altre, evidentemente, secondo alcuni intervenuti, risposte non soddisfacenti. Ma credo che sia un fatto davvero positivo. sicuramente non sono stati approvati emendamenti molto opportuni, che sollevavano ed offrivano proposte di soluzioni a problemi importanti,

un ambito limitato, per cui molti emendamenti sono stati colpiti da dichiarazioni di inammissibilità, dichiarazioni assolutamente ineccepibili, anche perché sono state formulate sulla base di criteri oggettivi che sono stati in tutti i casi applicati. Questo ci dice che sarebbe opportuno avere la possibilità, nel prosieguo dei lavori di questa legislatura, di affrontare molti di questi elementi in provvedimenti più ampi che non abbiano le limitazioni date da un decreto-legge (per di più un decreto-legge che verte sulla proroga dei termini), ovvero - perché no? - in provvedimenti di iniziativa parlamentare, che non devono necessariamente essere dei dei provvedimenti di decine e decine di articoli, che magari illustrano con la loro portata innovativa la persona del primo firmatario, per cui si può parlare della «legge Tizio» e della «legge Caio», ma possono essere piccoli provvedimenti che risolvono problemi importanti, che sollevano per esempio i cittadini da obblighi ormai non più motivati. Molte di queste cose sono state fatte, ed è davvero motivo di soddisfazione averle potute fare. Questo non vuol dire che non ci siano stati molti scontenti in merito a determinati emendamenti, ma questo è lo scopo del Parlamento: confrontare le varie opinioni, le varie posizioni. Vorrei sottolineare un punto importante: quello della proroga di certe materie per quanto riguarda l'entrata in vigore, l'inizio dell'istituto della mediazione previsto dalla riforma della giustizia civile

nell'affermare che è stata fatta quantomeno una forzatura (lui si è espresso in modo molto più forte) per quanto riguarda l'approvazione degli emendamenti (sono state due modifiche quelle apportate alla disciplina della mediazione), ha omesso un fatto molto importante, e cioè che nel corso della nel corso della discussione erano stati accantonati ben 19 emendamenti su questo argomento e che per un fraintendimento non era stato accantonato l'emendamento a firma, appunto, del senatore Lusi e di diversi altri colleghi che si limitava ad intervenire sui termini termini entro i quali sarebbe entrato in vigore l'istituto della mediazione. Questo emendamento comunque è stato approvato, la sua portata è stata pienamente rispettata, perché vi è una proroga di 12 mesi nell'entrata in vigore di questo nuovo istituto, ma gli altri 19 emendamenti che erano stati accantonati con l'intento di accantonare tutta la materia per trattarla unitariamente e per dare maggiore organicità e maggiore ordine alla discussione ve ne erano numerosi che ve ne erano numerosi che chiedevano la limitazione della proroga ad alcune materie. Questo è stato sintetizzato in un emendamento dei relatori e il combinato disposto dei due emendamenti (quello del senatore Lusi, che ha ritardato di 12 mesi l'entrata in vigore di questo istituto, e quello dei relatori, che ha limitato la proroga a determinate materie) ha rispecchiato pienamente la volontà della Commissione. Questo, anche perché certamente il secondo emendamento è stato votato nella piena consapevolezza di consapevolezza di come si combinava con quello approvato inizialmente. Pertanto, trovo spiacevole essere accusati di aver fatto una forzatura, quando semmai la forzatura è stata quella di non chiedere l'accantonamento anche di quel primo emendamento, che verteva sulla medesima materia sulla quale si era chiesto l'accantonamento per tutte le altre proposte provenienti dai senatori. Desidero precisare, con riferimento a quanto riferito dalla collega Spadoni Urbani a proposito dell'intervento che è stato fatto per la questione edilizia della Campania, che c'era, sì, una proposta di riapertura dei termini del condono edilizio, ma non è questa la proposta che è stata approvata. È stata approvata, infatti, una dell'entrata in vigore dei provvedimenti di demolizione per alcuni edifici della Campania, proroga che abbiamo ritenuto opportuno approvare in quanto in Campania, a differenza di tutte le altre Regioni, non era stato possibile applicare il condono edilizio del 2003: quindi è esattamente l'opposto. Qualcuno ha anche detto qui - non ricordo chi, forse un collega dell'opposizione - che solo in Campania vengono rinviati provvedimenti di demolizione, cosa che, invece, non avviene in nessun altra Regione d'Italia. Sarebbe stato più aderente al vero dire che solo in Campania, nel 2003, non è stato possibile presentare l'istanza

con due distinti provvedimenti, entrambi giudicati illegittimi dalla Corte costituzionale, aveva disapplicato in quella Regione un provvedimento che era legge dello Stato in tutte le altre Regioni d'Italia. Pertanto, è esattamente il contrario: è un equiparare la Regione Campania alle altre. Naturalmente, coloro che erano contrari al condono edilizio nel 2003 continueranno ad esserlo oggi, ma di fronte a una disparità palese tra gli abitanti della Campania e quelli delle altre Regioni credo che occorrerebbe una visione Le colleghe senatrici Bastico e Germontani hanno lamentato una scarsa chiarezza normativa nel testo di questo provvedimento. È un problema che credo credo tutti i parlamentari abbiano ben presente, non solo quelli che si trovano ad avere a che fare con la legislazione del nostro Paese, tanto che due anni fa fu approvato un disegno di legge governativo che comprendeva molte altre norme, in particolare un articolo che solennemente prevedeva

dovesse essere esplicitata la materia alla quale ogni provvedimento si riferisce. Questo, al fine di evitare le cosiddette norme mute, che sono, almeno a prima vista,

di diversi Governi, ma messo in atto sotto questo Governo: mi riferisco, cioè, a quel portale informatico «Normattiva» che ci permette di consultare le leggi con grandissima facilità. Tuttavia, le norme mute implicano ancora una consultazione.

Più che appellarsi al Governo affinché metta in atto quanto previsto da una legge, peraltro dallo stesso Governo proposta, oggi non possiamo fare. Va detto che spesso anche leggi di iniziativa parlamentare non rispettano questo dettato rivolto al Governo, che sarebbe bene fosse assunto come proprio anche dai parlamentari nelle loro iniziative o di disegni di legge o di emendamenti.

assistita. In ogni caso, anche fuori da quest'Aula si è molto parlato della trasmissione dei dati da parte delle strutture sanitarie che praticano la procreazione medicalmente assistita al Ministero

e non può esserlo, indipendentemente dalla volontà di chi ha presentato l'emendamento, poiché la legge vale per quello che essa reca, e non per le intenzioni di chi ha scritto la singola norma. In nessuno modo questa trasmissione di dati essere interpretata nel senso di creare quella cosiddetta schedatura delle donne di cui molti esponenti politici si sono fatti avversari ed hanno denunciato. Non può esserlo, perché la norma che abbiamo approvato in Commissione non prevede un'eccezione rispetto alla legge sulla

e non può certo essere superata per il fatto che in una certa norma si parla di trasmissione di dati. Poiché è chiaro che la trasmissione al Ministero dei dati riguardanti la procreazione medicalmente assistita serve unicamente per un un controllo dal punto di vista delle procedure e dei risultati di tale pratica, che è disciplinata da una legge relativamente recente, mi sembra perfettamente normale che il Ministero della salute voglia avere un quadro d'insieme per capire quali sono i risultati, quali sono le procedure che vengono seguite, anche perché non in tutte le Regioni...

il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, testé citato dalla collega - di controllare l'efficacia delle procedure e il rispetto delle normative vigenti.

il fondo destinato al 5 per mille, cioè alle scelte che liberamente e singolarmente possono fare i contribuenti per la destinazione di una quota dell'imposta

io non ho mai firmato, come Capogruppo nella Commissione giustizia, e nemmeno i colleghi della Commissione stessa lo hanno fatto, alcun emendamento che volesse limitare il rinvio dell'entrata in vigore della media conciliazione soltanto ad alcune materie e non ad altre, ma esclusivamente il rinvio complessivo

Innanzitutto, volendo chiarire, non è un provvedimento di riforma, né un disegno di cambiamento epocale: è un provvedimento che ha, come fine, proroghe di legislazione vigente, in alcuni casi fino al 31 dicembre, quindi con intervallo intermedio, in altri con scadenze ravvicinate, anche se, ed stato colto,

del Patto di stabilità, che è il rompicapo a cui l'Europa - per fortuna - ci lega e che si ribalta sulla realtà degli enti locali.

discussione che c'è da sempre tra i bilancisti. Se si raggruppano le poste di bilancio per macroaree c'è una maggiore flessibilità del bilancio, una maggiore possibilità per il Governo di collocare le poste sulle leggi

ferma restando la possibilità per il Parlamento di dare gli indirizzi. Come ho detto, scelte ci sono state, anche da parte del Governo e della maggioranza. Il caso di BancoPosta è una, ma molte altre sono state elencate nel dibattito. L'ultima considerazione generale è che proprio nel chiedere la riforma, molti interventi hanno richiamato il Consiglio europeo di marzo. Effettivamente noi siamo alla vigilia di una data epocale. È giusto che il Parlamento colga ogni occasione per porre l'accento su questo tema che ci impegnerà da domani: si determineranno probabilmente le nuove regole e anche

Agli studenti va il saluto dell'Assemblea.

poche considerazioni in sede di replica, dopo questa discussione su un provvedimento fortemente dibattuto, ma ad avviso del Governo significativamente migliorato e con elementi sicuramente discussi in Commissione ma che hanno apportato nuovi strumenti di disponibilità per poter affrontare questa congiuntura e questa fase così complessa da parte del Paese.

relativamente a precedenti conversioni di decreti di medesima materia, possiamo tranquillamente rilevare che, proprio di fronte alla mole così ingente di emendamenti (1.800), le modifiche apportate dalla Commissione sono sostanzialmente in media rispetto alle modifiche degli anni precedenti: sono circa un centinaio le modifiche; l'anno scorso sono state, se non ricordo male, circa 90. Ho dato questo numero, apparentemente banale, per dire che invece l'attività del Senato, delle due Commissioni riunite è stata assolutamente responsabile, puntando prioritariamente a modifiche virtuose del testo che prevedessero, come materia principale (se andiamo a vedere la natura delle modifiche degli emendamenti approvati), sostanzialmente proroghe di termini, e anche alcune questioni, come sempre accade peraltro di fronte ad un decreto decreto di materia eterogenea, con una parte prevalente quale quella della proroga di termini normativi, ma che tradizionalmente affronta alcuni temi del Paese, che sono di sostanziale congiuntura.

in una logica *bipartisan,* tra gli interventi sostanzialmente condivisi di questa legislatura, una riforma della legge di contabilità e di bilancio, che ha prodotto degli esiti che consideriamo assolutamente positivi, riguardanti prioritariamente il ciclo e ovviamente la sessione di bilancio, in particolar modo la legge di stabilità, ma che ha asciugato la possibilità per il Parlamento di presentare proposte emendative che ovviamente tengano conto delle sollecitazioni provenienti dal territorio, degli stimoli che vengono dal Paese e che hanno raramente occasione, all'interno di provvedimenti in fase di conversione, di poter essere affrontati. È evidente che molti di questi elementi hanno sostanzialmente natura di impatto economico e che è molto più difficile, ormai, rappresentare queste istanze nelle leggi di stabilità, queste giuste pulsioni si sono scaricate nel dibattito e nella presentazione così cospicua di emendamenti al provvedimento di proroga dei termini. Credo che in questo non ci sia nulla di scandaloso: è un atto di dialogo tra maggioranza e opposizione su questi argomenti. E credo che il Governo si sia presentato più che mai a questo appuntamento con un'assoluta disponibilità a valutare nel merito le proposte di modifica e a cercare di accogliere il maggior numero possibile di quelle fra alle due caratteristiche cui facevo prima riferimento: la prima, la proroga dei termini; la seconda, elementi di priorità considerati come tali nell'agenda della congiuntura del Paese. del Paese. Se andiamo a vedere la natura degli interventi, c'è stato, credo, un passaggio importante, su cui il Governo ha dato pieno assenso, tra gli elementi di contestazione: il fatto che si togliesse indisponibilità, sostanzialmente, alla norma primaria, l'elemento prioritario della proroga di termini, assegnandolo ad un decreto che possa essere attuato da parte della Presidenza del Consiglio relativamente alle proroghe successive a quelle in scadenza

rispetto a un'esigenza che ha ravvisato anche il Governo. Nel momento in cui si rinvia ad uno strumento non di rango primario l'eventuale proroga, è evidente, infatti, che si vuole togliere dall'arena

sarebbe stato più utile, più corretto ed anche costituzionalmente più adeguato intervenire per una modifica, riportando l'attenzione a questo passaggio in sede parlamentare. Si tratta pertanto di una modifica che noi consideriamo assolutamente virtuosa,

che sono andati ad affrontare temi che ovviamente sono vitali nella società del Paese. Non voglio qui ricordarli tutti, ma credo che alcuni di essi meritino una particolare attenzione per ribadire come questo provvedimento sia stato comunque un provvedimento virtuoso. Un primo argomento è quello della spesa. Come spesso può capitare, di fronte a segnalazioni e a emendamenti che rispondono anche a logiche di rappresentatività del territorio, il rischio è che ci possa essere un esito finale di

ha avuto un orientamento chiarissimo, che è stato quello di destinare alcune risorse a sensibilità di carattere parlamentare, come è stato evidenziato. Su di esse ovviamente è sempre possibile opinare, opinare, perché individuare le priorità rispetto a realtà che operano nel Paese o all'estero individuando le risorse da destinare, specie se poche

in realtà in cui ci sono delle priorità che comunque dovevano essere affrontate e che, pur nella logica del risparmio di spesa complessiva, dei cosiddetti tagli, evidentemente hanno a volte necessità di reintegro. una parte significativa di interventi riguarda, per esempio, il Patto di stabilità, poco ricordato in questa sede. Uno degli argomenti su cui oggi c'è un dibattito fortissimo nel Paese concerne l'attuazione progressiva dei decreti sul federalismo fiscale,

per consentire nei prossimi mesi una gestione meno rigida del Patto di stabilità, mantenendo comunque gli obiettivi virtuosi di bilancio e di controllo della spesa che ci siamo dati. Allo stesso tempo, abbiamo lavorato per mettere le Regioni nelle condizioni di affrontare altri argomenti, quali il tema della spesa sanitaria e quindi del Patto della salute. Sicuramente, in questo tipo di logica, uno degli elementi che ha suscitato molto dibattito ha riguardato la possibilità per i presidenti delle Regioni di intervenire sull'aspetto dei tributi e

Possiamo discutere o meno, come è stato fatto in questa sede, dell'opportunità di un'assunzione di responsabilità da parte dei territori, in particolar modo di quelli vicini a coloro che hanno subito questi eventi calamitosi, ma credo che il principio della responsabilità sia un elemento da cui non possiamo più prescindere nel momento in cui ci sono eventi di natura emergenziale e calamitosa che colpiscono questi territori, che devono prevedere sicuramente una solidarietà nazionale ampia ma anche una responsabilizzazione

delle iniziative di carattere internazionale per salvaguardarsi dalla fase congiunturale di crisi che stiamo attraversando. È di queste ore il dibattito e - pare - la chiusura dell'accordo in sede internazionale sulle risorse del cosiddetto fondo di stabilità e di salvaguardia degli Stati, che dovrà far fronte a quelli che sono stati eventi assolutamente negativi nei confronti dei bilanci di alcuni dei Paesi, Grecia *in primis* ma anche che si stanno ovviamente affrontando in sede europea. Gli interventi che abbiamo portato avanti con una serie di norme di proroga e di successivi emendamenti in questa sede consentono all'Italia di mantenere nei prossimi giorni un profilo alto e di continuare quindi ad affrontare tale argomento con grande determinazione e con la credibilità che ci siamo anche ritagliati rispetto a conti pubblici che sono in sostanziale sicurezza e che danno una prospettiva di tenuta al sistema Paese per i prossimi mesi.

comunque impegnate in termini di investimento per consentire a tali fondazioni di mantenere un patrimonio significativo nel tempo e quindi avere la possibilità di intervenire ulteriormente a sostegno di iniziative sul territorio, ma anche una serie di altri interventi di natura fiscale

al raggiungimento degli obiettivi: 25 miliardi di entrate, un record straordinario di lotta evidente all'evasione.

dare la possibilità al contribuente di poter onorare il proprio impegno, il proprio debito, nel rapporto con l'autorità e con il fisco in modo molto più concreto

il Parlamento*. Signor Presidente, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento 1.900, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2518, di conversione in legge del decreto-legge decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

e siamo convinti che lei recepirà questa nostra sollecitazione - un'applicazione attenta e puntuale del nostro Regolamento in riferimento al vaglio di ammissibilità degli emendamenti. Ciò, anche alla luce del parere della Giunta per il Regolamento reso l'8 novembre 1984, in cui si sanciva che: «in sede di conversione di un decreto-legge, la norma del primo comma dell'articolo 97 del Regolamento secondo la quale non sono proponibili emendamenti che siano estranei all'oggetto della discussione -» (e da notizie di corridoio pare ci sia nuova materia rispetto a quanto già esaminato) «deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche della indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78 del Regolamento, con riferimento sia al decreto-legge che al disegno di legge di conversione». Il richiamo al parere della Giunta di una verifica particolarmente rigorosa è ovviamente giustificato dalla notizia che si tratta di un maxiemendamento totalmente sostitutivo. Già la norma che noi stavamo esaminando aveva un contenuto eterogeneo, ora viene ad essere sostituita. Quindi, Presidente, le chiediamo veramente, per il rispetto del Parlamento, del Senato - e lei presta molta cura al rispetto della nostra istituzione - di verificare che non vengano stravolte le regole parlamentari, vanificando

si è discusso più volte in Conferenza dei Capigruppo dell'andamento dei lavori relativi a questo decreto-legge abbastanza impegnativo, di varia portata, diversamente dai decreti milleproroghe del passato, e che si è convenuto con la sollecitazione di questa Presidenza sul fatto che il testo del maxiemendamento eventuale rispecchiasse il lavoro della Commissione. Verificheremo questo, ma le posso assicurare di aver esercitato in questi giorni la mia attività di controllo affinché questa intesa venisse rispettata, pur non avendo naturalmente elementi procedurali che mi potessero portare ad impedire al Governo l'inserimento di parti nuove. Vi è un tema particolarmente delicato che è stato introdotto, che credo sia noto a tutte le parti, di maggioranza e di opposizione, che è quello relativo ad una norma attinente attinente alla tutela del sistema bancario, per il quale la 5a Commissione si è riunita, informalmente ieri, e stamattina formalmente, per dare un parere consultivo, dato che ormai non era più in sede referente. Un passaggio, questo, stimolato da questa Presidenza per fare in modo che nuovi argomenti di significativa portata potessero vedere nuovamente coinvolta la Commissione competente. Così è stato, e mi risulta che, stamani, la 5a Commissione ha lavorato a lungo su questo testo. È evidente che, se nel maxiemendamento dovessero, nelle parti eventualmente nuove, esserci degli argomenti totalmente estranei alla materia, che comunque - le posso assicurare - è molto ampia, eserciteremo la nostra vigilanza.

al testo dell'emendamento sia stata presentata la relazione tecnica. Altrimenti, il deferimento dell'emendamento alla Commissione bilancio da lei disposto non potrebbe dar luogo alla riunione, perché non sapremmo cosa giudicare.

convocazione che dispongo immediatamente, ma rientra nell'autogestione della Commissione. Anche questa Presidenza auspica che vi sia la relazione tecnica per consentirvi di realizzare opportunamente e compiutamente i vostri lavori di controllo.

dal Resoconto che ho avuto modo di leggere ho rinvenuto delle cose francamente inesatte che il relatore Malan ha riferito, e siccome mi cita personalmente, e la cosa mi riguarda personalmente, chiedo la cortesia di poter fare una precisazione. Il relatore Malan, in ordine ad una questione già nota a coloro che se ne sono occupati durante lo svolgimento dei lavori delle Commissioni riunite, ha riferito in Aula che io avrei omesso nel mio intervento di ieri un fatto molto importante, cioè che nel corso della discussione erano stati accantonati ben 19 emendamenti su questo argomento - media conciliazione - e che per un fraintendimento non era stato accantonato l'emendamento a firma mia (e, ricordo al relatore Malan e agli altri colleghi, di moltissimi altri colleghi di tutti i Gruppi parlamentari) riguardante appunto il rinvio dell'applicazione dell'istituto della media conciliazione. Signor Presidente, è doveroso che io ricordi due questioni. Non si è mai visto un senatore che, dopo che il Governo e il relatore hanno dato parere favorevole, chieda l'accantonamento dell'emendamento. Non l'ho mai visto in vita mia; forse mi mancava, nella mia esperienza personale. Né tantomeno ho mai visto che due Commissioni riunite che votano all'unanimità un emendamento possano essere tacciate di aver omesso qualcosa. In secondo luogo, signor Presidente, si è parlato di un emendamento 1.316 (testo 2) che recherebbe la mia firma e quella di molti altri colleghi. Ripeto qui, perché sia messo a verbale, che né il sottoscritto né gli altri colleghi che risultano in questo fantomatico emendamento 1.316 (testo 2) hanno mai né sottoscritto né depositato un testo 2 dell'emendamento 1.316. L'unico testo che noi abbiamo depositato e sottoscritto è l'emendamento 1.316, sottoposto all'approvazione delle Commissioni riunite e approvato all'unanimità. il senatore Malan omette di ricordare nella sua replica, purtroppo poco puntuale da questo punto di vista, è che quello che lui chiama fraintendimento io non lo giudico in modo diverso, ma c'è stata su questo tema una violazione del procedimento legislativo. Ho provato a spiegarlo ieri, in modo calmo e tranquillo, non omettendo alcun passaggio di ciò che è avvenuto nelle Commissioni riunite. L'ordine di radicalità con il quale l'emendamento del relatore è stato presentato - emendamento che ha modificato la norma come veniva producendosi a valle dell'emendamento di rinvio 1.316 - ha violato il procedimento legislativo, perché l'emendamento del relatore era meno radicale di quello che era stato votato nei giorni precedenti nelle Commissioni riunite. In questo senso, quell'emendamento era e doveva essere dichiarato inammissibile. Su questo tema, mi rendo conto

di fronte ad un errore, se di errore si trattava, nella gestione dei pareri da parte della maggioranza. Non si è voluto trovare e si è dato uno schiaffo. Il risultato, a lei non distante - e ho concluso, signor Presidente - è che l'effetto prodotto, a dimostrazione del fatto che quello che abbiamo affermato è corretto, è che il combinato disposto degli emendamenti approvati in sede di Commissioni riunite, l'1.316 e quello del relatore, approvato 24 ore dopo, è che la norma entri in vigore prima della legislazione attualmente vigente, a conferma che il procedimento legislativo è stato palesemente e patentemente viziato.

disperate, che non ce la fanno più ad arrivare alla fine del mese, andate a salvare le banche e gli interessi dei banchieri! Spero che sia stata ritirata la norma

però, in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, la norma di cui all'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. c'è una sentenza delle sezioni unite della Cassazione civile del 2 dicembre del 2010 che ha stabilito che tutti gli imprenditori che sono stati «usurati» dall'anatocismo bancario, ossia dagli interessi sugli interessi,

io continuo a difendere i diritti della povera gente ma voi, cari membri del Governo, continuate a difendere gli interessi dei banchieri. Mi auguro che si vada presto al voto, perché la gente non ce la fa più. La Corte di cassazione fa le sentenze e voi le disfate, come la tela di Penelope. Sono davvero indignato, e mi scuserà, signor Presidente, di ciò. La ringrazio molto per avermi dato la parola, però davvero non ci sono parole:

L'emendamento 1.316, sappiamo bene, ha avuto un solo testo: questo testo è stato approvato, è stato rispettato nel successivo andamento dei lavori ed è incluso nel maxiemendamento. Pertanto, credo sarebbe ora di smetterla con tale questione, perché è stata

che non hanno fatto o di aver menzionato testi 2 che non hanno menzionato*.

in relazione a richieste di alcuni Gruppi di opposizione. Le dichiarazioni di voto avranno inizio intorno alle ore 19. Seguirà quindi la chiama sulla fiducia, intorno alle ore 20. Nella seduta antimeridiana di domani avrà inizio la discussione del decreto-legge recante proroga di missioni internazionali. Nel pomeriggio di domani, alle ore 16, il Ministro degli affari esteri renderà un'informativa sui più recenti sviluppi della situazione nei Paesi del Mediterraneo. Seguirà un'informativa del Governo sugli sbarchi di clandestini a Lampedusa. Su entrambi gli argomenti i Gruppi potranno intervenire rispettivamente per cinque minuti ciascuno. Nel corso di questa settimana, ove concluso dalla Commissione, sarà anche discusso il disegno di legge sulla parità di accesso nei consigli di amministrazione. Il calendario della settimana corrente è stato integrato con lo svolgimento di interpellanze e interrogazioni, che avrà luogo nel corso della seduta antimeridiana di giovedì 17 febbraio. Pertanto, le già previste sedute pomeridiana di giovedì 17 e antimeridiana di venerdì 18 non avranno luogo. La prossima settimana, nella seduta pomeridiana di martedì 22 febbraio e nella seduta antimeridiana di mercoledì 23 si svolgerà la discussione sulle comunicazioni del Governo sullo schema di decreto legislativo in materia di federalismo municipale, con eventuale voto di proposte di risoluzione. Sempre nel corso della prossima settimana si procederà all'eventuale seguito del richiamato disegno di legge sulla parità di accesso, nonché alla discussione del disegno di legge sui prodotti ortofrutticoli di quarta gamma e della mozione Scanu sul poligono militare di Quirra.